nei mesi scorsi diverse associazioni di categoria del settore cerealicolo hanno manifestato in piazza per denunciare il crollo dei prezzi, in particolare del grano. L'offerta di cereali italiani non trova infatti collocazione sul mercato, se non con grande difficoltà, poiché i nostri cereali risultano economicamente meno competitivi di quelli prodotti in altri Paesi europei, che utilizzano *standard* produttivi diversi e controlli qualitativi meno rigidi rispetto ai nostri. in pericolo non solo la produzione di grano e la sopravvivenza di oltre 300.000 aziende agricole che lo coltivano, ma anche un territorio - specie nel Sud d'Italia - di due milioni di ettari a rischio desertificazione, ma soprattutto gli alti livelli qualitativi per i consumatori garantiti dalla produzione *made in Italy*. Da pochi centesimi al chilo concessi agli agricoltori dipende la sopravvivenza della filiera più rappresentativa del *made in Italy*, mentre dal grano alla pasta i prezzi aumentano di circa il 500 per cento e quelli dal grano al pane addirittura del 1.400 per cento. Quali misure il Governo intende adottare per regolare il mercato? Qual è lo stato di realizzazione delle misure previste dall'accordo siglato al Ministero lo scorso 20 luglio con le organizzazioni sindacali e istituzionali del settore cerealicolo? Quali iniziative sono state prese per dare forza alla filiera grano-pane-pasta italiani? In particolare, non da ultimo, quante risorse sono state previste nella legge di stabilità o in ulteriori provvedimenti per incrementare il fondo, attualmente di 10 milioni, così come annunciato dallo stesso Governo, che sappiamo essere interessato in maniera piena a che questa filiera cresca e si rafforzi?

a circa 10 milioni di euro. Sono decisamente un'inezia rispetto al problema. Se li dovessimo dividere per tutti i quintali prodotti, facendo i classici conti molto banali, ma chiari

interventi di carattere estemporaneo e non programmatico, nemmeno di tutela rispetto a elementi legati a eventi imprevisti, come aethina tumida e xylella. Certo si capisce come ci sia una direzione che vada verso il miglioramento della produttività del settore attraverso nuove tecnologie, ma la fotografia che emerge fa il paio con l'ultimo *report* annuario sull'agricoltura. Mi spiego meglio: dai dati presenti nell'analisi dell'annuario, il settore agricolo risulterebbe in crescita. Andando più nello specifico, però, aumenta il consumo di suolo, il comparto che potremmo definire classico è in sostanziale stagnazione, come ci dicono gli agricoltori, mentre il settore che cresce di più è quello legato all'impiantistica di smaltimento a biomassa e a biogas,

ci sono problemi analoghi. Soffermiamoci innanzitutto sul settore dei cereali. Il Governo ha già preso qualche provvedimento: ha istituito il Fondo per le imprese cerealicole e mi sembra che questo vada nella giusta direzione, con l'obiettivo di sostenere i contratti di filiera, di valorizzare la qualità, di incentivare l'uso di sementi certificate e il marchio unico volontario. La dotazione però, Ministro, andrebbe certamente aumentata: lo intendo come un primo stanziamento. Bisogna sostenere i nostri produttori e credere in loro

una Commissione unica per il grano duro e l'annunciato strumento assicurativo di garanzia: sarebbe bene che lei facesse il punto su questi strumenti.

dunque, il Ministero in questa direzione? Non è il caso di porre mano, con energia, all'elaborazione di un piano strategico nazionale, evidentemente in accordo con le categorie interessate? Signor Ministro, diamo un segno di speranza concreta ai nostri produttori.

è, nel nostro Paese, il più importante luogo di transito e scarico di grano importato, proveniente per la maggior parte da Turchia, Ucraina e Canada.

Di fatto, quindi, quello che sempre più si manifestava come un deterrente, sebbene debole e non sempre efficace, perché non associato ad una politica di sostegno adeguata, è stato definitivamente tolto di mezzo. Attualmente, secondo la Coldiretti, in Italia un pacco di pasta su cinque è già prodotto interamente con grano canadese. A questi dati aggiungo la disposizione del Ministero della salute sul divieto in Italia dell'uso del glifosato

come il grano proveniente da USA e Canada, dove viene fatto un uso intensivo di questo e di altri erbicidi proprio nella fase di pre-raccolta, per seccare e garantire artificialmente un livello proteico elevato. Le chiedo quindi, signor Ministro, attraverso quali iniziative intende far fronte a quello che rischia di diventare un vero *tsunami* giallo sul nostro Paese.

ad esempio l'accordo con il Marocco, ai fini della liberalizzazione reciproca dei prodotti agricoli, tra cui i pomodori, che possono quindi essere esportati con dazi molto bassi alle frontiere italiane. Tali accordi stanno dunque aggravando ulteriormente la crisi che colpisce un settore molto rilevante della nostra economia ortofrutticola. considerare, ancora, che le medesime violazioni della concorrenza e la mancanza di una efficace tracciabilità e reale trasparenza nei confronti dei consumatori stanno avvenendo anche nel settore del grano, che l'Italia importa in quantità significative, 4,8 milioni di tonnellate di grano tenero e 2,3 milioni di tonnellate di grano duro, e che la legislazione europea non prevede alcun obbligo di indicare la provenienza del grano sull'etichetta, con il risultato che, pur acquistando marchi italiani, il consumatore non può accertarsi che per la loro produzione sia stato utilizzato grano *made in Italy*. Alla luce di queste considerazioni, si chiede di sapere: in che modo il signor Ministro intenda promuovere adeguate misure di sostegno alle aziende che operano nel settore ortofrutticolo, ai fini del ripristino di una effettiva competitività; se intende attivarsi con sollecitudine, presso le opportune sedi, al fine di adottare misure volte a prevedere un maggior rigore nelle procedure di controllo degli *standard* igienici e sanitari sui prodotti ortofrutticoli importati, soprattutto dal Nord Africa; quali iniziative intenda assumere, nelle opportune sedi europee, per tutelare gli interessi del settore cerealicolo e ortofrutticolo nazionale e se non creda necessario inaugurare occasioni di confronto con le Regioni meridionali maggiormente interessate.

Ciò significa che siamo arrivati veramente all'estremo. Oggi chiedere ai nostri agricoltori di continuare su questa china, quando abbiamo un'importazione e una concorrenza straniera che manda fuori mercato la produzione di frumento italiano, significa chiedere di rinunciare alla propria tra attività, perché il costo è ormai Sappiamo e, purtroppo, siamo ormai consapevoli, che siamo arrivati sotto i 18 euro al quintale per i produttori agricoli, che non riescono nemmeno a coprire i costi di produzione, contro i 180 euro al quintale pagati dai consumatori per la pasta secca prodotta. A questo punto chiediamo al Ministro quali iniziative serie, reali e concrete si stanno mettendo in conto e si stanno facendo, perché non può più essere semplicemente una dichiarazione di principio, bisogna che si passi veramente ai fatti e i fatti necessitano di misure anche nei confronti di dazi e nei confronti di provvedimenti che blocchino l'importazione straniera. LIUZZI *(CoR)*. Signor Ministro, i settori cerealicolo e ortofrutticolo sono pesantemente indeboliti dalla concorrenza selvaggia e dalla diseguaglianza fiscale e contributiva dei nostri diretti concorrenti europei e mediterranei. Come s'intendono valorizzare le nostre produzioni e tutelare la continuità reddituale e la piena occupazione del settore? Di recente, il Governo, con il legittimo e giusto intento di contrastare il caporalato, ha di fatto inflitto nuovi e maggiori oneri ed adempimenti complessi al settore, che rischiano però di mettere in ginocchio l'intero comprato ortofrutticolo. In che maniera si intende intervenire onde evitare la definitiva chiusura di migliaia di aziende con la perdita di miliardi di euro di fatturato e, soprattutto, di migliaia di posti di lavoro? In relazione al settore cerealicolo assistiamo ad una vergognosa speculazione che vede i nostri agricoltori fallire e i truffatori internazionali arricchirsi. Come si intende intervenire? In che maniera il Governo potrebbe valutare la possibilità di utilizzare prioritariamente il grano duro prodotto nel nostro Paese e, successivamente, quello proveniente dall'estero. In Puglia, signor Ministro, ci sono esempi virtuosi in tal senso, eccellenze di pastifici che producono e trasformano grano proveniente dai territori contermini pugliese e lucano. C'è un piano di concerto con le organizzazioni categoriali e agricole che preveda e valorizzi la filiera del grano e della pasta e che privilegi il prodotto interamente *made in Italy*?

abbiamo iniziato a lavorare sull'idea di un piano nazionale per la filiera grano-pasta, con la consapevolezza che anche questa filiera, come - ahimè - altre filiere agroalimentari del nostro Paese, vivono un *deficit* organizzativo interno che ereditiamo da una situazione oggettivamente fragile degli anni passati che in qualche modo noi dobbiamo oggi cercare di superare. Concretamente, per la prima volta questo Paese si dota di un piano nazionale cerealicolo con 10 milioni di euro come prima posta di bilancio per attivare alcuni strumenti. Sono assolutamente d'accordo con voi che non sono sufficienti, ma bisogna lavorare affinché

tuttavia, che questa prima posta di bilancio ha consentito nelle settimane scorse di iniziare un'attività, in particolare sui contratti di filiera, per accompagnare un lavoro unitario di produttori e trasformatori in alcuni territori, al fine di aiutare ad uscire dalla complicata in cui eravamo nelle settimane scorse. Già oggi i prezzi sono diversi da quelli di qualche settimana fa, il che non vuol dire, ovviamente, che abbiamo risolto tutto il tema, ma siamo certamente di fronte a uno scenario migliore, su cui impostare una strategia. Non c'è alcun dubbio che una delle leve su cui vogliamo investire è proprio quella dei contratti di filiera, con l'obiettivo di incrementare gli ettari a contratto di filiera in questo Paese. Siamo a 80.000 ettari; possiamo arrivare, ragionevolmente, in tempi rapidi, a 100.000 ettari se spingiamo attraverso questi meccanismi, quindi se dotiamo il produttore e il trasformatore, che siglano un contratto d'intesa sulla qualità, sulle quantità e sul prezzo, di un*quid* in più determinato dal contributo che possiamo offrire noi. Quei 100 euro a ettaro che noi oggi mettiamo sul contratto di filiera non risolvono interamente la questione, ma sono una variabile non indifferente per consentire un utilizzo sensibile di questi contratti. Le reazioni che ci sono sui territori più interessati - penso all'Emilia-Romagna, alla Puglia, alle grandi Regioni cerealicole in particolare, in Puglia dimostrano che gli effetti di questo nuovo strumento si stanno facendo sentire e secondo me sono una premessa del lavoro che dobbiamo fare. fare. Oltre a questo, segnalo che, a proposito di fondi europei, abbiamo confermato nel luglio scorso, proprio nel pieno della crisi crisi di mercato, aiuti accoppiati europei (PAC) per il frumento per un equivalente di 70 milioni di euro l'anno per i prossimi sette anni. Potete facilmente fare il conto: ci stiamo sostanzialmente impegnando con la filiera, in particolare con gli aiuti accoppiati, per un intervento che è di quasi 500 milioni nei prossimi sette anni. Sono aiuti accoppiati che vanno direttamente al produttore e sono una parte di quella integrazione che garantiamo nel medio lungo periodo, in particolare per l'anello più debole della filiera. Il terzo aspetto è stato richiamato dal presidente Formigoni ed è uno dei temi per me più rilevanti. Siamo nelle condizioni, prima della prossima campagna, di poter sperimentare, unici in Europa, un'assicurazione sui ricavi proprio per i produttori di grano. Abbiamo lavorato all'impalcatura fondamentale dello strumento assicurativo

capiremo se, effettivamente, con l'assicurazione riusciremo a contribuire, nei momenti più difficili del mercato, a sostenere, in particolare, i produttori. Sostanzialmente, abbiamo definito i fondamentali di questo lavoro sulle polizze all'interno del piano assicurativo agricolo annuale. Voglio citare un ultimo punto su questo fronte, cruciale per noi: siamo nelle condizioni ormai, d'intesa con il ministro Calenda, di fare un passo storico sul versante della tracciabilità e dell'etichettatura. Esattamente nel solco del lavoro svolto con il latte, saremo nelle condizioni, nelle prossime giornate, di chiudere una sperimentazione italiana di tracciabilità ed etichettatura della filiera grano‑pasta che segnerà un punto, a mio giudizio, di svolta, dopo tante discussioni negli anni rispetto a questa questione. Ci stiamo lavorando con il Ministero dello sviluppo economico e, devo dire in un rapporto molto positivo, con tutta la filiera, e credo che questo sarà un punto fondamentale per garantire gli elementi, richiamati anche da voi, di maggiore informazione, tracciabilità e riconoscibilità del prodotto nella filiera grano-pasta. Per quanto riguarda intanto un cappello generale. Se siamo arrivati fin qui con una operazione di forte riduzione della pressione fiscale, prima con l'abolizione dell'IMU, poi con l'abolizione dell'IRAP, infine con l'abolizione dell'IRPEF agricola in questa manovra di bilancio, queste scelte non sono state avventate o estemporanee, ma rispondono a un argomento fondamentale, che abbiamo sempre avuto in testa: tutelare il reddito di chi vive di agricoltura con tutte le leve possibili; la leva fiscale per un Governo è una delle più immediate. L'abbassamento della pressione fiscale con il superamento di queste tre imposte segna un punto di svolta notevole per un comparto. Molto concretamente, stiamo parlando di un miliardo e 300 milioni in meno di tasse in due anni. Non è tutto, vi è ancora molto da fare, ma è senz'altro una scelta che, a mio avviso, ha una portata a suo modo storica, visto come il come il comparto era stato fin qui gestito e trattato. Sul fronte dell'ortofrutta, è chiaro che il tema fondamentale è quello organizzativo. Noi abbiamo la gigantesca necessità di lavorare di più e meglio sulle organizzazioni dei produttori. In tante realtà dove andiamo in crisi quando il mercato fa fatica, il primo vero argomento è la disorganizzazione dei produttori. Bisogna dirlo in maniera chiara. Non è possibile, in alcune realtà, avere una molteplicità di soggetti che da soli non riescono a reggere le crisi di mercato. Tutte le vere esperienze di tenuta nella crisi le abbiamo anche nel settore dell'ortofrutta, quando le organizzazioni dei produttori sono strutturate in obiettivo è quello di lavorare di più, d'intesa con la filiera, alla riorganizzazione delle regole per la costituzione e la promozione delle organizzazioni dei produttori. produttori. Noi abbiamo l'occasione della nuova strategia nazionale per l'OCM ortofrutta che, lo segnalo, in questo Paese è sempre stata gestita e utilizzata molto bene. molto bene. Quello è lo strumento forte per fare questo salto di qualità tutto organizzativo, perché senza questo cambio di passo non ci sarà nessuno strumento per gestire una dinamica di mercato che ha delle complessità stagionali perfino indefinibili da anno ad anno e che varia, spesso, da settimana a settimana. Questa è la leva vera su cui stiamo cercando di insistere. Aggiungo anche che, invece, per quanto riguarda

milioni dedicati ad alcuni lavori molto specifici, specificamente alle colture *made in Italy* dei nostri territori, sono un fatto di assoluta rilevanza che non si vedeva da tempo. Questo Piano si interseca anche con la grande novità di Industria 4.0, dove abbiamo lavorato, sempre insieme al ministro Calenda e al MISE, a uno specifico investimento sul versante dell'agricoltura di precisione come asse di sviluppo fondamentale per il comparto primario. Il fatto che questi due percorsi possano viaggiare di pari passo per me segna una occasione straordinaria per fare in modo che si sviluppino innovazione e tecnologia sul versante delle nostre colture *made in Italy*, andando - e lo vedrete nel piano ricerca - coltura per coltura, ad indicare precisamente dove investiamo, per quale ragione, verso quale obiettivo. Siamo nelle condizioni, con il Piano, di fare questo salto di qualità. Lo presenteremo, nello specifico, nei prossimi giorni all'Accademia dei Georgofili a Firenze e io ritengo che si potrà vedere, anche in successivi passi di confronto parlamentare, che questo Piano accompagna una scommessa di innovazione

RUTA *(PD)*. Signor Ministro, bene i contratti di filiera; bene l'azione sulle assicurazioni; bene l'intesa con il MISE per l'etichetta narrante di cui l'Italia ha bisogno: gli italiani, i consumatori, non solo il mercato interno, ma anche quello estero. Sul *made in Italy* noi giochiamo il nostro futuro. Quindi, su un tipo di agricoltura e non solo su una qualunque agricoltura. Per questo già siamo il Paese più controllato e per questo la direzione è quella giusta. Resta il problema finanziario,

oltre che da senatore, sono seriamente preoccupato. Signor Ministro, non è così che risolviamo i problemi della nostra agricoltura, se a un certo punto ci adeguiamo anche alle norme europee sull'etichettatura e accettiamo che venga tolto, sull'olio di oliva, il luogo di produzione del prodotto.

progetti di studio sulle centrali a biogas che sono alimentate da cereali di bassa qualità; non le ho chiesto se le piaceva il programma che ha presentato, perché immagino che le piaccia. Infatti, se lei dà incentivi alle centrali a biogas e mette soldi per studiare il compostaggio anaerobico per produrre energia, è chiaro che va verso la produzione di

A me piacerebbe, ogni volta che viene in Aula, che studiasse la risposta alle domande e non faccia uno *show* su quello che produce. Va bene la ricerca, va bene l'agricoltura di precisione, ma non era questa la domanda. La domanda era: come avete potuto incentivare le centrali a biogas che utilizzano cereali di bassa qualità anziché potenziare il *made in Italy* di qualità.

Certamente i nostri agricoltori si trovano di fronte a difficoltà tradizionali che sono state incrementate dalla terribile crisi economica che tutti conosciamo, ma il Governo e il Parlamento si sono mossi nella giusta direzione. Oggi lei ha assunto impegni importanti, che tutti noi teniamo a mente e sottolineiamo, perché bisogna andare avanti nel sostenere un settore che in questi anni, nonostante le difficoltà, ha saputo crescere ha fatto in maniera molto significativa. Per cui aumentiamo gli stanziamenti e andiamo verso quel nuovo contratto di assicurazione del reddito, perché queste sono le strade che l'agricoltura moderna insegna e di fronte alle quali gli operatori italiani sapranno reagire positivamente.

immaginavo che ci prospettasse le iniziative che il Governo intende adottare da oggi in avanti e non ci raccontasse le iniziative che sono già state adottate e che appaiono, alla luce dei risultati, quantomeno da un punto di vista quantitativo, insoddisfacenti. Mi auguro che da questo punto di vista ci sia un cambio di passo, poiché anche le buone intenzioni, quelle del piano cerealicolo o di una sperimentazione del progetto sulla tracciabilità, per essere interpretate al meglio hanno bisogno di un'assistenza finanziaria. Infatti un piano cerealicolo per un Paese come l'Italia con una dotazione di 10 milioni su due anni diventa soltanto un manifesto e nulla di più. E noi, purtroppo, non abbiamo bisogno di manifesti, ma di intervenire con forza su problemi che ormai sono diventati strutturali.

Ministro, nel suo intervento si è fatto vanto di una tracciabilità e di una filiera che invece hanno bisogno di molta più concretezza;

estrema dipendenza dalle volontà e dalle scelte dell'Unione europea. Su questi aspetti vogliamo molta più determinazione rispetto a quella che il Governo sta dimostrando e non si può lasciare un risultato al silenzio-assenso, devono esser fatte delle affermazioni.

rispetto alla validità del nostro impegno sui tavoli che contano in Europa nei decenni trascorsi, di cui oggi facciamo ancora le spese. Avrei Avrei desiderato che il Ministro mi dicesse qualcosa di più preciso in merito alla lotta al caporalato e in particolare all'intento di non criminalizzare tutte le aziende che fanno ancora il loro dovere in campo agricolo.

È importante perché ritengo che lavorare per aumentare la salubrità delle produzioni, migliorare la qualità dei terreni, garantire la tracciabilità produttiva e ridurre i tempi improduttivi aumentando la redditività delle imprese significhi lavorare per consolidare i fattori fondamentali per la competitività del settore agricolo italiano.

Di forte impatto per l'incremento di innovazioni tecnologiche sarà il Piano industria 4.0 che, oltre ad avere una impostazione giustamente intersettoriale e una gestione interministeriale, prevede un sistema di incentivazioni decisivo per un'accelerazione dell'impiego di tecnologie e attrezzature meccaniche. Si chiede quindi di sapere qual è lo stato dell'arte della programmazione dell'agricoltura di precisione e Agrifood prevista all'interno del Piano industria 4.0 visto che il piano prevede la possibilità di aumentare l'ammortamento fino al 250 per cento anche per le macchine agricole, se sono state individuate dalla commissione appositamente le tipologie in dettaglio delle macchine agricole che potranno beneficiare dell'iperammortamento, che porterebbe ad un risparmio fino al 36 per cento e dunque ad una reale opportunità

e così importante se non si sommano più effetti contemporaneamente. Pertanto, non possiamo puntare solo sull'agricoltura di precisione, migliorando le tecniche, le tecnologie, il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente,

All'inizio dell'anno lei, signor Ministro, si è dichiarato contro gli OGM e devo apprezzare molto l'*optout* che ha firmato per non coltivarli sul territorio nazionale. Tuttavia, lei ha finanziato la ricerca sulle nuove biotecnologie che, secondo tutto il mondo scientifico, sono comunque OGM e quindi vanno trattate con estrema cautela, tant'è che abbiamo chiesto e ottenuto, qui in Senato, Senato, un affare assegnato, proprio per valutare l'impatto, la brevettualità e la proprietà intellettuale di queste nuove biotecnologie per renderle fruibili e democratiche sul territorio nazionale e soprattutto prive di rischio. Trovo adesso, nell'atto di riordino del CREA per il triennio 2017-2019, in fase di valutazione il progetto sul post-Expo, per il quale il centro ha avanzato una proposta che si chiama «Seed development and seed composition: genetic bases and effects on human health». che lo Human technopole sarà una *partnership* pubblico-privata e noi siamo particolarmente preoccupati dal colosso Bayer Monsanto, che preoccupa non solo noi, ma anche gli addetti alla ricerca pubblica, che temono di non essere in grado di competere con questi colossi. Vorrei capire se nello Human technopole ci sarà effettivamente una *partnership* pubblico-privata per questi nuovi *seed development* e, se sì, quali tutele state mettendo in atto per evitare che la ricerca pubblica sia sopraffatta da questi colossi che, usciti dalla porta, rientrano dalla finestra e abbattono qualunque speranza di un «*made in»* e di un miglioramento genetico di qualità, che sia approvato da tutte le associazioni agricole, dai movimenti e dalle

perché devono affrontare molteplici e difficili problematiche, alcune immediate e alcune future, quali la progressiva diminuzione delle risorse energetiche e primarie attualmente utilizzate (petrolio e acqua su tutte), il costante aumento dei prezzi per l'acquisto dei fattori produttivi, la diminuzione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, l'inquinamento ambientale, il benessere animale e il continuo e inarrestabile mutamento del clima. Prima dell'arrivo dei macchinari e dei concimi di sintesi - i cosiddetti concimi chimici - l'agricoltura tradizionale aveva una produttività molto bassa. Gli anni Duemila hanno visto il picco produttivo proprio grazie ai combustibili fossili. In un futuro prossimo, però, sarà obbligo praticare, con il minor utilizzo possibile di energia fossile, una zootecnia e un'agricoltura ad alto grado di sostenibilità che, allo stesso tempo, siano capaci di sfamare la popolazione mondiale. Dunque, l'innovazione tecnologica è fondamentale, come lo è stata nel passaggio dal lavoro manuale a quello meccanico e dal lavoro meccanico a quello più intellettuale. L'incremento delle tecnologie innovative (quindi l'automazione e il maggior utilizzo dei sistemi informativi come GPS, GIS e VRT), inducono miglioramenti importantissimi in campo operativo (più *hardware*) e direttivo (più *software*). Alcuni esempi sono la guida assistita e automatica delle macchine agricole, l'eliminazione delle rilavorazioni e delle sovrapposizioni, la misura precisa delle produzioni, il monitoraggio dello stato del terreno e delle colture tramite sensori, così da poter regolare le lavorazioni e organizzare distribuzioni differenziate. Si chiede pertanto al signor Ministro se in tali ambiti non sia necessario fornire incentivi, di diversa natura, affinché le aziende si possano dotare delle tecnologie più recenti, al fine di incrementare, nell'ambito di un'agricoltura di precisione, l'attività produttiva, rendendola, al contempo, più sostenibile in secondo luogo, se non sia necessario favorire una maggiore diffusione delle conoscenze e delle ricerche in tali settori, mettendo a disposizione delle aziende una rete di supporti altamente qualificati e indipendenti (CREA, università) per

La maggior parte di tali sistemi opera mediante un ricevitore GPS collegato al trattore agricolo o alla mietitrebbiatrice, permettendo l'identificazione in tempo reale della posizione, con la conseguenza, per esempio, di agire direttamente sullo sterzo dove il GPS mantiene esattamente parallele le passate, apportando come benefici un minore *stress* per l'operatore, risparmio di tempo e di sprechi perché evita le sovrapposizioni. Sfruttando sempre sistemi GPS è possibile localizzare *a posteriori* il luogo esatto dove si era prelevato un campione del terreno da analizzare. Inoltre, esistono sistemi che possono rilevare i diversi parametri delle produzioni in campo. È importante consultare tali dati per capire in quali zone si è prodotto di più e in quali meno, e perché: questo aiuta nelle scelte da effettuare nell'anno seguente. Alla luce, quindi, dell'importanza che gli strumenti di innovazione tecnologica assumono per i nostri agricoltori, si chiede di sapere se il signor Ministro non ritenga opportuno che il Governo preveda taluni incentivi, anche nella forma della detrazione fiscale, per quegli agricoltori che vorranno elaborare nella loro azienda strategie

Signor Ministro, credo che per dare un senso a questo nostro *question time* si possa, sì, parlare di agricoltura di precisione e di introduzione di strumenti innovativi e tecnologia, come è stato concordato, ma non si può far finta che la situazione per l'agricoltura nelle zone

Stiamo parlando di un'area che dà al nostro Paese notorietà, fatturato e orgoglio di produzione. Stiamo parlando di persone che fanno agricoltura in maniera anche eroica, restando sui monti quando molti altri giovani, oggi, se ne sarebbero già andati.

una copertura alle stalle crollate, piuttosto che interventi di copertura agli stessi agricoltori: una roulotte, un camper, un modo per poter rimanere vicino ai propri allevamenti, alle proprie attività produttive, alle proprie stalle. Già da queste cose si dà l'idea di un Paese che ha l'orgoglio della propria produzione e della propria attività agricola. Le chiedo anche, Ministro, insieme alla Commissione o altrimenti, di fare un'azione di verifica sul territorio di persona:

Riscontriamo finalmente un processo virtuoso che va incoraggiato da parte del Governo, da parte, cioè, di chi detiene le leve del potere e quindi può decidere insieme al Parlamento, alle Regioni, e d'intesa con l'Unione europea. Questo fenomeno virtuoso riguarda i giovani e il loro convinto ritorno all'agricoltura, al settore primario per antonomasia. I giovani non vanno delusi e nemmeno illusi. propongono quali nuovi alfieri dello sviluppo sostenibile, che si fonda sull'uso massiccio di tecnologia, dalle nanotecnologie alle biotecnologie, come pure le *information and communications technology*. Essi vanno collocati in filiera con i centri di ricerca e le università italiane ed estere, cioè con i centri del sapere che sanno trasferire competenze. L'agricoltura meccanizzata ha rappresentato un traguardo raggiunto nella seconda metà del Novecento. È giunta l'ora della informatizzazione in agricoltura, dell'agricoltura informatizzata che investa i settori dell'ortofrutta, della cerealicoltura, dell'allevamento e dell'industria casearia. Il Governo come intende intervenire in tal senso? In che maniera intende promuovere la cooperazione tra enti, università e centri di ricerca? In che maniera si intende intervenire per promuovere l'impegno di giovani e di figure specializzate in grado di rafforzare la qualità delle risorse umane? In che maniera, infine, l'utilizzo di strumenti di precisione possono trovare riscontro nelle informazioni a disposizione dei consumatori?

È vero che il fronte agricolo è estremamente delicato: siamo passati in un colpo da circa 300 imprese coinvolte dal sisma del 24 agosto a 3.000 imprese agricole coinvolte, secondo una prima stima ancora non completa. Si può quindi capire la complessità dell'intervento. Stiamo lavorando alacremente. Posso confermare che nella giornata dell'altro ieri,

ad animale, per dare immediatamente un sostegno agli allevatori e garantire la continuità aziendale in una condizione estremamente delicata. Per poter garantire la continuità c'è bisogno di un intervento il più rapido possibile con strutture temporanee per far questo, verranno raddoppiate immediatamente le quantità sia di stalle temporanee che di alloggi abitativi temporanei dedicati agli agricoltori.

che abbiamo già pagato per 29.000 imprese agricole di quei territori (sostanzialmente, tutte le imprese agricole delle Province coinvolte) 65 milioni di euro di contributi agricoli, tutti in un'unica soluzione per

al tema di un aggancio diretto al settore agricolo. Si sono citati i GPS come soluzioni tecnologiche per il settore: c'è una casistica precisa di strumentazioni che sono inserite nelle schede tecniche del Piano industria 4.0 e quindi possono usufruire dello strumento del superammortamento. Non escluderei un ampliamento di queste tecnologie, attraverso una fase emendativa, che possiamo sviluppare insieme, mentre rafforziamo questo Piano, perché credo che questa sia la leva vera che abbiamo per intensificare il lavoro e arrivare all'obbiettivo del 10 per cento di superficie. Aggiungo che siamo in fase di definizione e di chiusura del bando INAIL sulla sicurezza e sull'innovazione della meccanica agricola,

ha una connessione giusta con la ricerca in campo agricolo e agroalimentare, perché tanta parte di questo lavoro si può sviluppare certamente anche sul versante

del progetto di ricerca sono saldamente in mano pubblica (e ci mancherebbe altro) e stiamo cercando di fare esattamente quello che fanno tanti altri Paesi nel mondo e da tempo.

cui un grande progetto come questo necessita, anche *step by step*, fase per fase. Siamo ancora nella fase di implementazione, di inizio di questo lavoro ed è di queste ore la notizia di una consistente finanziamento pubblico del Governo sul progetto del *campus* universitario dell'Università statale di Milano che integrerà il progetto dello Human technopole, che credo rilevi

dallo spazio pubblico, in autonomia, con grande professionalità, come si fa sempre quando si cerca di svolgere un lavoro di avanzamento efficace,

faticoso impegno di progettazione verrà definita compiuta ed inizieranno i primi passi di Human Technopole. Torno a dire, e chiudo, che ritengo si sia di fronte ad un'occasione, l'occasione di provare a far fare al nostro Paese, in particolare al modello agricolo italiano, un salto di qualità significativo proprio sul versante delle tecnologie e dell'innovazione. Abbiamo in giro delle belle esperienze che in questi anni hanno praticato innovazione, senza aspettare lo Stato;

di interventi che da tempo il nostro Paese aspettava. quanto riguarda le zone colpite dal sisma, stiamo seguendo direttamente il suo lavoro insieme alle Regioni e lo apprezziamo. Tornando al tema del *question time*, esprimo soddisfazione per gli obiettivi e il percorso che lei ci ha indicato. Abbiamo la consapevolezza che scegliendo di investire sull'agricoltura di precisione, in realtà, si sceglie un nuovo concetto e un nuovo approccio per l'agricoltura: più tecnologie, meno chimica, più efficienza, più

che vanno affrontati seriamente. Mi meraviglio di quella legge appena approvata da questo Parlamento, dal Parlamento italiano: si dice no agli OGM e poi si consente la libera circolazione dei prodotti all'interno del nostro Paese incontrollatamente e deliberatamente. Cominciamo a lavorare su questi temi seriamente, senza queste discrepanze.

mi sembra di capire che in realtà non state facendo alcun tipo di strutturazione per evitare che tutta questa ricerca vada a cadere poi nel settore privatistico, mentre le assicuro che dall'indagine conoscitiva che stiamo conducendo in Senato emerge questo rischio.

rassicurare sulla distribuzione delle risorse, sul reale collegamento tra centri di potere e centri della ricerca a disposizione dell'agricoltura e sulla necessità di tenere